per usare un termine asettico – interessanti innovazioni nel nostro sistema giuridico e processualpenale, e quindi richiede la giusta e doverosa attenzione.

Siamo molto preoccupati e credo che anche a nome dell’intero Parlamento possiamo estendere i sentimenti di vicinanza ai familiari e di preoccupazione per la sua sorte, che ci auguriamo sia seguita con particolare attenzione anche dalla Farnesina, non soltanto da Emergency. Ma la riflessione che vogliamo lasciare al Parlamento e` di un’estrema preoccupazione per alcuni termini che, anche se non confermati poi nella sostanza, sono stati espressi e che oggi trovano spazio sulla stampa. In particolare, ci sarebbe la richiesta, da parte di un gruppo di tagliagole, della consegna di un cittadino che ha ottenuto asilo politico in Italia,

qualche volta cosı` sconsiderate, nei confronti delle richieste del mondo islamico. (Applausi

Presidente, spero che non sia semplicemente un rito quello che compiamo in queste fasi della seduta.

Intervengo per sollecitare una presa di posizione sua e del Senato che faccia seguito ad una ancora piuautorevole, perche´ proviene dal Quirinale,

in nome di non si sa bene quale inopportunita. L’articolo 21 della Costituzione sancisce la libertadi pensiero e credo che in questo Paese anche il diritto di scrivere verita scomode vada rispettato.

polemiche e persino in accordi internazionali fra Paesi sul revisionismo nei libri di testo. Persino questo accade tra Cina e Corea o tra Giappone e Cina. Che in questo Paese uno scrittore voglia scrivere quello che ritiene e informare e informare i cittadini di avere svolto opera di ricerca nella storia e questo possa fargli rischiare fisicamente il diritto di esprimere le proprie idee credo sia un fatto grave. Apprezzo

Assemblea debba esprimere massima solidarieta` a Giampaolo Pansa perche´ in questo Paese si deve essere liberi di poter esprimere le proprie idee senza che gruppi di teppisti possano impedirlo.

Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Storace, Storace, essendo un lettore abituale degli scritti e dei libri di Pansa, che nell’ultimo periodo nelle sue opere approfondisce elementi dibattuti della nostra storia recente,

enorme questione. Mi consenta di dire che non la risolveremo – ahime! – con il dibattito in Aula, anche se ha un grande rilievo. Se si deve aspettare qualche giorno in piu,